Informo altresì l'Assemblea che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 17 ottobre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha indicate valide: per Regione Trentino-Alto Adige: Michaela Biancofiore, Meinhard Durnwalder, Pietro Patton, Luigi Spagnolli, Elena Testor e Julia Unterberger. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni. una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 novembre. Nella seduta di oggi si terrà la discussione generale del decreto-legge in materia di qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Il seguito dell'esame del provvedimento, fino alla sua conclusione, avrà luogo nella seduta di domani, per la quale è previsto l'orario di chiusura alle ore 14. La prossima settimana l'Assemblea si riunirà a partire da martedì 24 ottobre, alle ore 14, fino a venerdì 27, se necessario, con sedute senza orario di chiusura. Oltre agli argomenti già previsti in calendario, sarà discusso il disegno di legge sulla competitività dei capitali, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al disegno di legge dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 19 ottobre. Il calendario prevede inoltre le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove presentato in tempo utile. Si ricorda inoltre che il calendario potrà essere integrato con il Rendiconto 2022 e il Bilancio interno 2023 del Senato. La settimana dal 30 ottobre al 2 novembre è riservata ai lavori delle Commissioni; l'Assemblea si riunirà solo per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi. Nella settimana dal 7 al 9 novembre saranno discussi i seguenti argomenti: disegni di legge istitutivi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sull'emergenza SARS-Cov-2 e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori; decreto-legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali; decreto-legge sulle politiche di coesione e immigrazione, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

e di biossido di azoto, che coinvolgono le medesime Regioni. L'articolo 1, comma 1, introduce dunque per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna l'obbligo di aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i provvedimenti attuativi alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti e di quanto previsto dal successivo comma 2. Durante l'esame in Commissione, anche alla luce di quanto evidenziato da alcuni dei soggetti auditi, il termine per l'aggiornamento è stato esteso da sei a dodici mesi. Nelle more dell'aggiornamento dei piani, il comma 2 stabilisce che le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, anche delle altre vetture e dei veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria N1, N2 e N3 che rientrino nella categoria euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone presso le quali risultano superati uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto. Durante l'esame in Commissione è stato specificato che le limitazioni alla circolazione stradale debbano essere strutturali e che le relative deroghe debbano essere motivate. A decorrere dal 1° ottobre 2025 la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 è inserita nei piani di qualità dell'area delle Regioni che adottano i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, autorizza le Regioni di cui al comma 1 a esentare dalle limitazioni alla circolazione autovetture e veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria euro 3 *monofuel* e *bifuel* alimentati con carburanti alternativi. Il comma 2-*ter*, anch'esso introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che, con decreto del Ministro Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria Durante l'esame in Commissione sono poi stati inseriti nel testo due articoli aggiuntivi. L'articolo 1-*bis* è volto ad incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione preservazione degli ecosistemi locali. A tal fine esso istituisce un fondo destinato al finanziamento di progetti e iniziative volte alla creazione e alla riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea ai fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea e in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'articolo 1-*ter* riconosce quale opera strategica di preminente interesse nazionale con carattere di indifferibilità,

oggi discutiamo è un decreto che si è reso necessario perché la Corte di giustizia ha condannato alcune nostre Regioni per un fatto abbastanza grave, cioè il continuo sforamento dei valori di emissioni delle sostanze più pericolose che abbiamo nell'aria che respiriamo: PM10 e PM2.5 sono degli inquinanti nuovi che riescono a penetrare nei sistemi polmonare e cardiocircolatorio e sono causa delle malattie più gravi che si registrano nel nostro Paese - leucemie e tumori e tumori - che creano sicuramente drammi all'interno delle famiglie italiane. Si stima che l'inquinamento atmosferico sia causa di 70.000 morti premature nel nostro Paese, un dato assolutamente allarmante. Siamo quindi chiamati

i piani di qualità dell'aria a misure più stringenti, che potrebbero consentire una riduzione delle emissioni clima-inquinanti.

Parliamo di morti premature e quello che cerchiamo di fare oggi è applicare le soluzioni che comunque la scienza, le università e anche le industrie stanno maturando da tempo. Non ci dobbiamo inventare nulla di nuovo. La politica arriva spesso con decenni di ritardo.

gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento con un'unica misura, perché derivano da più determinanti. Ci sono sicuramente il trasporto nelle città, il riscaldamento e la questione legata all'agricoltura: queste determinanti hanno un elemento in comune, che è la combustione. Nel momento in cui incentiviamo sistemi che si basano sulla combustione di energie fossili,

disincentivare dal punto di vista economico, anche facendo cassa, tutto quello che è combustione. Noi dobbiamo, ad esempio, smettere di incentivare sistemi di riscaldamento basati sulla combustione, perché non hanno senso, che inquinano e si basano su fonti di energia che compriamo dall'estero. Dobbiamo invece incentivare sistemi di riscaldamento basati su fonti rinnovabili che produciamo in Italia e su sistemi che non prevedono la combustione, tipo le pompe di calore.

l'auto elettrica piace, ma perché ha un motore assolutamente più efficiente. Basti pensare che nel traffico di Roma un'auto a combustione interna ha un'efficienza del 7 per cento - ciò significa che è una stufa con quattro ruote, perché si tratta di motore endotermico, e maggiore l'effetto calore che l'effetto mobilità - mentre un'auto elettrica ha un'efficienza intorno al 96 per cento: è normale che il mercato andrà in quella direzione. Non ci sarà Ministro che fermerà questa evoluzione. Le vendite in Europa delle auto elettriche sono esplose, perché è la tecnologia che avanza e noi non potremo fare nulla per fermarla. È inutile che ci inventiamo un metodo per fermare questa tecnologia, perché sia le industrie, sia i centri di ricerca hanno già studiato modelli di sviluppo che consentono all'umanità, che cresce in maniera rilevante sul pianeta, di trovare sistemi che una qualità della vita elevata grazie alle fonti rinnovabili. Quindi cosa dobbiamo fare? Sostanzialmente abbiamo già tracciato dei disegni di legge in materia: abbiamo parlato di reddito energetico e un altro disegno di legge incentiva proprio le fonti non basate sulla combustione, come le pompe di calore, per cui chiediamo ad esempio una detrazione al 100 per cento, e il fotovoltaico, il solare termico, le piastre a induzione

una riduzione delle tasse deve essere non per tutti, ma solo per chi ha comportamenti virtuosi. Le vostre norme di legge sono tutte piatte e anche questo disegno di legge non produrrà effetti nei prossimi anni. Probabilmente l'inquinamento in quelle zone aumenterà, perché sono disegni piatti che non producono effetti. Invece dovreste pensare a disegni di legge che defiscalizzano tutto ciò che non è basato sulla combustione. Come Come riuscire poi a coprire il costo di questa defiscalizzazione? Si aumentano le tasse su quello su ciò che inquina, su ciò che è basato sulla combustione. Allora, in questo caso riuscite a trovare pareggio senza andare in *deficit*. Posso anche pensare di andare in *deficit* se faccio qualcosa di virtuoso, ma andare in *deficit* per abbassare di poco le tasse a tutti è qualcosa di assolutamente sbagliato che non serve in questo periodo storico. Noi possiamo andare in *deficit* se facciamo delle manovre virtuose, di contemperare tutte le esigenze che ci sono, quelle ambientali e quelle climatiche. Una manovra finanziaria piatta, che opera un piccolo taglio a tutti, non serve a nessuno

muoverci e riscaldare le nostre case in maniera sostenibile e con prezzi bassi per un medio-lungo periodo. *(Applausi)*. E questo lo possiamo fare con cosa?

Noi dobbiamo utilizzare l'energia che abbiamo. Siamo un Paese ricco e abbiamo molte più fonti da rinnovabili di quelle di cui abbiamo bisogno. Quindi, dobbiamo utilizzare queste fonti, che sono disponibili, a basso prezzo a basso prezzo e costano per i prossimi trent'anni, rendendole disponibili per tutti. E lo dobbiamo fare infischiandocene delle *lobby* che vogliono continuare a vendere caramente l'energia agli italiani. Noi non siamo il Governo delle *lobby* del petrolio e delle *lobby* del gas. *(Applausi)*. Noi siamo il Governo dei cittadini italiani. E, se siete il Governo dei cittadini italiani, dovete fare l'interesse dei cittadini e non delle *lobby* petrolifere e del gas, che hanno solo un interesse: vendere l'energia e realizzare magari extra profitti. Questo a noi non interessa. Dobbiamo fare una manovra che serva a tutti e serva soprattutto al popolo, ai cittadini italiani. L'unica manovra che può consentirci di diminuire i costi dell'energia e di diminuire l'inquinamento è utilizzare le fonti rinnovabili e fare un superbonus, magari con delle percentuali più basse, soprattutto per chi può investire.

se non le risana lo Stato, non le risana nessuno. Si devono lasciare almeno delle percentuali per gli alloggi popolari, per chi comunque vive in un edificio di proprietà statale, e l'unico modo è quello. se la calibriamo bene, non ha costi per lo Stato; se cioè la calibriamo facendo sì che ci siano delle entrate dovute a maggior occupazione, più posti di lavoro

accumulando, a comprare le nuove tecnologie dall'estero, perché stiamo perdendo il treno e purtroppo lo stiamo perdendo per colpa di questo Governo.

il provvedimento in esame oggi è un atto importante, che prosegue nel tentativo di arginare un problema risalente. Per apprezzare la bontà di questo decreto dobbiamo ricordare che la prima la prima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per il superamento sistematico e continuato dei valori limiti applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani, risale al 2014; superamento che in anni successivi viene constatato anche per il biossido di azoto. La norma prevede l'obbligo, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, di aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria e anche, se necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro sei mesi. Prevede anche uno slittamento della limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali *diesel* euro 5, sempre nel bacino padano, dal 1° ottobre 2024 nei centri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che siano ricadenti in zone nelle quali si è verificato il superamento di uno o più dei valori limite di materia inquinante. Questa limitazione diventa obbligatoria dal 1° ottobre 2025. Questo, quindi, in estrema sintesi è il contenuto del provvedimento in discussione oggi. Ora, gentili colleghi, vorrei portare alla vostra attenzione due questioni in particolare. La prima è l'urgenza della situazione, che ha bisogno di una risposta immediata e di una terapia d'urto. Ecco perché viene previsto il termine di soli sei mesi per l'aggiornamento, da parte delle Regioni, dei piani di qualità dell'aria. La seconda questione riguarda il problema della qualità dell'aria. È un problema multifattoriale e, come tale, necessita di un approccio sistemico e programmatico. Quanto alla questione dell'urgenza, è bene partire da una considerazione che non tema smentite: quello ambientale è un settore importante, un settore nel quale non ci dovrebbero essere opposizioni, perché ogni provvedimento che va che va nella direzione di migliorare le condizioni ambientali è uno strumento in più per tutelare la salute di questa generazione e soprattutto delle future. Non capisco quindi le critiche a questo provvedimento, se non attribuendole al solito ambientalismo ideologico, che è solo di facciata e non ha mai risolto i problemi. Ogni provvedimento è perfettibile, e lo dico con sincerità. E se ho imparato qualcosa quando ho svolto l'incarico di assessore all'ambiente della mia Regione, la Basilicata, è che, quando si parla di ambiente, si può fare sempre di meglio. Questo non vuole assolutamente dire che, in attesa di fare meglio, si debba rimanere immobili: tutt'altro. Non c'è ambito pubblico più soggetto ad emergenze di quello ambientale; e alle emergenze bisogna rispondere subito e con provvedimenti che possano dare nell'immediato risposte. Questo è un provvedimento emergenziale e le opposizioni che hanno governato fino a un anno fa dovrebbero saperlo meglio di tutti. *(Applausi)*. L'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia europea ben due volte, perché, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone ha superato i limiti delle particelle PM10 di biossido di azoto. La Corte ha riconosciuto una riduzione progressiva dei livelli di concentrazione e un miglioramento della qualità dell'aria, come hanno certificato anche l'ARPA Lombardia e l'Istituto superiore di sanità. Ma questo non è bastato a evitare le condanne. I livelli di PM10 di biossido d'azoto devono rimanere sotto i limiti. Il problema dello sforamento dei limiti previsti in Pianura padana, quindi, è più complesso di quanto si pensi. Tanto è confermato anche dall'Agenzia europea dell'ambiente che, nel suo ultimo *report* sullo stato della qualità dell'aria in Europa, relativo all'anno 2022, 2022, segnala tra le zone con i dati peggiori la nostra Pianura padana, definita area densamente popolata e industrializzata, con specifiche condizioni meteorologiche e geografiche che favoriscono l'accumulo di inquinanti dell'aria e nell'atmosfera. Questa definizione è la perfetta sintesi dei presupposti su cui poggia il provvedimento oggi in discussione. La Pianura padana è una delle aree più densamente popolate e più industrializzate d'Italia. Non si può pensare di mettere in crisi famiglie e imprese creando un enorme problema problema sociale, bloccando la circolazione dei veicoli *diesel* euro 5 già da quest'anno, anche in considerazione - così come emerge dalla relazione - della difficoltà di reperire i materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici. Per questo, il decreto-legge in discussione oggi sposta in avanti la data di applicazione delle misure di limitazione della circolazione per i veicoli di categoria *diesel* euro 5. Lo sposta avanti di un anno, in linea con gli obiettivi europei, come ha precisato più volte il ministro Pichetto Fratin. Anche con questo provvedimento, il Governo si dimostra di buon senso. Il termine viene spostato in avanti, ma viene data una accelerata all'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria delle Regioni del bacino padano, che la stessa norma individua come strumenti principali nel riportare i valori degli inquinanti al di sotto delle soglie consentite. Il piano di qualità dell'aria è, del resto, la fotografia delle caratteristiche del territorio, delle fonti di emissioni, degli inquinanti in aria, delle condizioni climatiche e meteorologiche e permette di individuare gli interventi ottimali per il risanamento. Qui arriviamo alla seconda questione che deve essere valutata parlando di questo provvedimento. La multifattorialità del problema qualità dell'aria può essere risolta solo attraverso più strumenti complementari, che incidano su tutte le cause di inquinamento, ma che devono essere inseriti in un quadro e in una programmazione coerente. A questo proposito dobbiamo ricordare che il primo accordo per il bacino padano risale al dicembre 2013 e individua tra i settori più inquinanti per l'atmosfera la conduzione di biomasse, il trasporto merci, quello passeggeri, il riscaldamento civile, l'industria, la produzione di energia e l'agricoltura. Il 9 giugno 2017 veniva sottoscritto dal ministro Galletti e dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un nuovo accordo di bacino padano per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria, che prevedeva azioni riguardanti tutti i settori suddetti. Dobbiamo ricordare anche che esiste già un fondo nazionale per l'attuazione di misure di miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano, istituito col decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Il fondo stanzia risorse fino al 2034 per misure relative ai trasporti e alla mobilità sostenibile, alla combustione domestica della biomassa e all'efficienza energetica, interessa anche il settore agricolo ed è stato incrementato da questo Governo con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 dal decreto-legge n. 13 del 2023. Anche sulla questione agricoltura sostenibile non dobbiamo dimenticare i provvedimenti che il ministro Lollobrigida ha confermato quali l'attivazione di risorse pari a 400 milioni di euro, previste nel PNRR, per lo sviluppo di macchinari agricoli a emissioni zero, cui si aggiungerà lo stanziamento di ulteriori 225 milioni a valere sul fondo per l'innovazione; ma potremmo citarne altri quali la prossima istituzione del registro CO2 o le misure per rendere il comparto dell'allevamento più sostenibile inserite nel piano strategico della PAC. È quindi ovvio che questo provvedimento è solo un ulteriore tassello per la soluzione del problema, con il quale si accelera sull'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria da un lato e, dall'altro, si cercano di calmierare le conseguenze della limitazione dei veicoli diesel euro 5, sempre nel rispetto degli obblighi europei; limitazione che, è inutile nascondercelo, avrà un impatto finanziario consistente ma giusto, come tutti i provvedimenti che mirano alla transizione ecologica, e che ricadrà sia sulle tasche dei cittadini che sulle finanze pubbliche e questo è un dato da non sottovalutare e da non sottacere, anche se le opposizioni tendono ad insabbiarlo. È un dato che i cittadini italiani devono tener presente quando si parla di conti pubblici. Diciamolo forte e chiaro: i conti pubblici sono strozzati, tra l'altro, dai venti miliardi di spese del superbonus. Non dobbiamo far finta di nulla, ma dobbiamo dire ai cittadini che quando qualche avvocato parla di provvedimenti gratis perché paga lo Stato e non gli italiani mente perché i cittadini sono lo Stato e se paga lo Stato pagano i cittadini. Questo si vede anche quando il Governo è costretto a fare una manovra asciutta e senza sprechi. Concludo dicendo che ancora una volta il Governo dimostra quella pragmaticità nelle scelte politiche che è indispensabile in situazioni che si trascinano da anni e che necessitano di soluzioni, senza dimenticare che queste si inseriscono in un panorama pianificatorio di più ampio respiro. Credo si possa affermare che è finita l'epoca dei provvedimenti *spot*, che tamponavano un problema senza porsi come obiettivo la soluzione. Sono sicuro che con questo provvedimento si darà un'accelerazione alla risoluzione ed al superamento dei limiti di inquinamento atmosferico ed esso sarà esso sarà determinante nel ripristino di un'ottimale qualità dell'aria nella pianura padana.

mira a dare esecuzione ad alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. più che un atto importante è un atto dovuto, perché senza l'adeguamento di questo piano della qualità dell'aria, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, a seguito delle procedure di infrazione di cui all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

quindi di una responsabilità non di questo Governo, ma di quelli precedenti. Io penso che se non usciamo da questa discussione, probabilmente non diamo un messaggio di verità a chi ci sta ascoltando. Il problema del livello del PM10 nelle aree della pianura padana, del Nord d'Italia, è un problema strutturale che dipende in parte dall'orografia, quindi dalla composizione del nostro territorio nazionale, e in parte da responsabilità che si sommano di Governo in Governo, di anno in anno. Come possiamo affrontare i temi? Innanzitutto capendo qual è il costo in termini di vite umane e il costo sociale che dobbiamo nel momento in cui non adottiamo misure di adattamento e mitigazione per la riduzione dei livelli di PM10. Finché non avremo chiaro qual è il costo della nostra mancanza di azione, è evidente che non avremo consapevolezza di quello che dobbiamo fare. Consentitemi di dire che questo decreto-legge è un compitino, è cioè ciò che dovevamo fare perché senza questo saremmo incorsi in una procedura di doppia condanna, ma è un'occasione mancata.

due opposte tentazioni. La prima è quella del negazionismo climatico di chi non riconosce che il tema del cambiamento climatico è una realtà e che il tema delle azioni di mitigazione e adattamento sono un dovere.

*(Applausi)*. Faccio qualche esempio concreto perché è giusto che noi lo sappiamo; in questo momento il ministro Pichetto Fratin è a Lussemburgo a chiedere la rinegoziazione di una direttiva che riguarda l'ETS marittimo, quindi non il tema alla nostra attenzione, ma una normativa per la quale se noi non riduciamo le emissioni di CO2 nel sistema del *transhipment* a livello globale, che senso ha obbligare i porti italiani ad adeguarsi a delle norme

si può pensare davvero di trovare una misura uguale per tutti i Paesi obbligando all'efficienza energetica del patrimonio edilizio. Certo, tutti noi vogliamo ridurre per esempio i consumi di CO2 nelle case, ma sappiamo perfettamente che abbiamo una differenza enorme rispetto al patrimonio abitativo degli altri Paesi. Signori, siamo l'Italia, un Paese che ha

Chi di noi non vorrebbe ridurre le emissioni di CO2 puntando sulle energie rinnovabili? Tutti, ma dobbiamo anche avere il coraggio di dire che non si può fare la transizione puntando solo sulle energie rinnovabili dall'oggi al domani perché il fabbisogno energetico del nostro Paese non può essere coperto integralmente dalle fonti rinnovabili. *(Applausi)*. Ciò significa diminuire la dipendenza energetica per esempio dal gas. E voi sapete quanto questo sia un tema non solo di competitività, ma anche di sicurezza internazionale, visto che noi dipendiamo principalmente da due Paesi: la Russia attraverso Gazprom e l'Algeria attraverso Sonatrach. Se non diminuiamo la dipendenza da poche fonti combustibili, è evidente che abbiamo anche problemi dal punto di vista geopolitico. Anche Anche alla luce di una votazione che c'è stata nel Parlamento europeo e di cui spesso facciamo finta di non cogliere le conseguenze qui nel Parlamento nazionale, credo che che, ad esempio, ripensare all'utilizzo del nucleare all'interno delle fonti *green* sia una di quelle questioni su cui il Parlamento deve cominciare a dire delle parole chiare. seguente. Se vogliamo diminuire il livello del PM10 in queste Regioni abbiamo bisogno di quella che si chiama cura del ferro:

la linea ferroviaria e alleggerendo le tangenziali che a volte sono realizzate vicino agli agglomerati urbani; significa che, piuttosto che penalizzare l'uso di questa o quella macchina, dovremmo capire che

interrompere l'utilizzo della macchina, posso favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale per arrivare alla mobilità dolce e a muoversi in maniera sostenibile all'interno delle città. Se noi non assumiamo il tema dell'intermodalità come chiave di lettura della mobilità, è evidente che rischiamo di nuovo di cadere nel tranello di chi non vuole cambiare il suo comportamento e di chi pensa che dall'oggi al domani basta seguire la sostenibilità per obbligare a muoversi in maniera sostenibile. Ci sono persone che purtroppo non possono farlo o per questioni economiche o per questioni di poca accessibilità accessibilità e di poca mobilità. Ecco perché, signor Presidente, spero che questa, che è una misura necessaria per non incorrere in una procedura di infrazione, non sia l'ennesima occasione in cui in cui prendiamo atto di ciò che è dovuto senza riflettere su ciò che avremmo dovuto fare e anche oggi perdiamo l'occasione di fare.

non stiamo facendo nient'altro. Vogliamo inoltre allungare i tempi su tutto quello che bisogna fare oggi per la qualità dell'aria e per ridurre le emissioni in aria? Sicuramente facciamolo, però il Governo - lo posso ribadire da questi banchi - e noi di Forza Italia siamo impegnati anche grazie al nostro Ministro dell'ambiente, che è sempre

quelle azioni necessarie soprattutto per migliorare la qualità dell'aria. Ma quelle sono anche aree produttive importanti, quindi bisogna coniugare varie esigenze per non bloccare il Paese. È giusto oggi ridurre l'inquinamento, però occorre fare attenzione perché parliamo della Pianura padana, che è un'area produttiva importante

di azoto, i cui livelli certamente devono essere monitorati. Non mancano - e sono anche a disposizione - le risorse economiche e finanziarie, pari a circa 90 milioni di euro per quest'anno e per gli anni successivi. Tali risorse servono al rafforzamento anche di soluzioni alternative di trasporto: se uno non può utilizzare Altre risorse importanti sono destinate al fondo nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano,

arrivare a inquinamento zero nel 2050. Peraltro, abbiamo invece un *target* intermedio al 2030, per cui bisogna ridurre comunque drasticamente gli agenti inquinanti. Dobbiamo quindi arrivare a che

va alla relatrice del provvedimento, la collega Petrucci, come anche al Presidente dell'8a Commissione, che ha lavorato su questo decreto fino a qualche minuto fa, e al nostro collega Claudio Fazzone, che hanno messo in campo una serie di emendamenti che hanno migliorato il testo, a dimostrazione

cari colleghi, dopo tanti decreti *omnibus* ci troviamo a votarne uno che si compone di un solo articolo. Se questo non è sintomo di perdurante bulimia da necessità e urgenza, sinceramente non saprei come definirla.

Non voglio però sembrare disfattista o eccessivamente di parte a questa Assemblea e ammetto che i provvedimenti fin qui varati dal Governo Meloni, compreso quest'ultimo, sono accomunati da un unico merito; hanno, per così dire, un minimo comune denominatore: qualcosa, infatti, ci dicono del livello di considerazione che questo Governo ha per la Costituzione, per il Parlamento e per le prerogative di tutti noi parlamentari. una mortificazione continua del ruolo e delle funzioni delle due Camere, che ha trovato recente conferma anche nelle gravissime

che la maggioranza evitasse di presentare emendamenti alla legge di bilancio. Si tratta di affermazioni aberranti che mi consentono, a questo punto, di consigliare al ministro Giorgetti di prendere l'esempio dall'abilissima e più scaltra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che riesce a farsi fissare all'ultimo minuto un appuntamento in agenda proprio a ridosso di una conferenza stampa, così da fuggire alle domande scomode dei giornalisti.

permette alla maggioranza di mettere una pezza, ma consentitemi di dire che questa pezza è peggio del buco, perché in buona sostanza non fate altro che perdere tempo ben sapendo che tempo da perdere non c'è n'è e che le risposte sarebbero dovute essere ben altre. Giovi a questa Assemblea ricordare che il decreto-legge qualità dell'aria è stato adottato in risposta a due sentenze della Corte di giustizia europea. Per farla breve, il nostro Paese è venuto meno agli obblighi previsti dalla direttiva unionale sulla qualità dell'aria anche a causa del mancato rispetto sistematico e continuativo del valore limite annuale fissato per il biossido d'azoto in alcune

Manca una visione consapevole e responsabile, soprattutto, del futuro della mobilità del nostro Paese. Manca una seria programmazione strategica di medio e lungo periodo. Si interviene quindi in maniera insufficiente sulla qualità dell'aria, concentrandosi esclusivamente sulle emissioni derivanti dalla circolazione stradale, senza affrontare la questione in maniera più ampia, ovvero tenendo conto anche delle emissioni connesse, ad esempio, alle attività agricole e zootecniche, agli allevamenti intensivi e alla presenza di termovalorizzatori, come giustamente ricordava la collega Sironi in Commissione. Non solo: voi e solo voi stabilite chi potrà circolare l'anno prossimo per le strade di queste Regioni, senza dirci nulla sulle opzioni di trasporto alternative che possono di fatto consentire ai cittadini di lasciare l'auto sotto casa. Voi e solo voi stabilite queste cose senza intervenire, ad esempio, con misure risolutive in agricoltura e negli allevamenti per limitare le emissioni dell'ammoniaca. E lo fate senza affrontare il tema cruciale del potenziamento delle infrastrutture su ferro, per traslare i trasporti dalla gomma al ferro. Colleghi della maggioranza, ora immagino che vi starete chiedendo: cosa si aspettava questa qui da un decreto che ha un solo articolo? Certo, nulla di più di quello che avete fatto. Ormai vi conosco, vi conosciamo, non potevamo aspettarci di più; potevate forse decidere una cosa, quella sì, vista la sostanziale insufficienza dei contenuti. Potevate decidere di inserire queste norme in uno dei tanti decreti *omnibus* che tanto vi piacciono. Questo decreto non dà risposte, al contrario pone ingombranti interrogativi proprio sulla vostra capacità di dare risposte. D'altra parte, c'è da comprendere il disagio che molti di voi certamente avvertiranno nel votare un mini decreto sulla qualità dell'aria, visto che due Ministri di questo Governo non fanno altro che parlare di quanto sia brutto l'elettrico, di quanto siano belli i termovalorizzatori e di quanto sia necessario il nucleare di nuova generazione che non esiste. fritta. Colleghi della maggioranza, per voi transizione ecologica ed energetica sono inutili orpelli. Non ci aspettavamo proposte concrete in questo provvedimento. Sappiamo benissimo come la pensate lo dico senza alcun tipo di pregiudizio verso alcuna forza politica qui rappresentata. Ma la domanda che mi faccio è la seguente: che Paese vogliamo essere? L'Italia può davvero permettersi di perdere tempo e restare indietro su temi tanto importanti, guardando passarsi avanti altri Paesi che sono pronti ad accettare nuove condizioni a sviluppare situazioni economiche maggiormente favorevoli per il proprio Paese? Possiamo permetterci di non programmare un avvenire sostenibile per il nostro Paese? Ancora, possiamo permetterci una classe politica ostinatamente inconsapevole e sorda in maniera allarmante su questioni tanto delicate, questioni che sono e saranno di certo alla base di qualsivoglia agenda politica che guardi al domani e che parli di futuro? Bene, la risposta è chiaramente inserita in questo decreto: per voi sì, questo si può fare. Bene, fatelo, ma non in nostro nome.

collega Di Girolamo, così come lo siamo della manovra che è stata approvata. Una manovra che non vi aspettavate e che vi ha spiazzato: dall'aumento delle pensioni agli stipendi minimi, al taglio del canone Rai e finalmente - la cosa che forse vi ha più spiazzati - la copertura del finanziamento del ponte sullo Stretto. Questo è un disegno di legge con cui vogliamo intervenire e con cui il Governo interviene con misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e delle conseguenti limitazioni della circolazione stradale. Con questa norma si intendono valorizzare i risultati ottenuti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente nel 2017, per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. È proprio nell'ambito di questo accordo di programma che le Regioni interessate hanno messo in campo interventi importanti intesi a migliorare la qualità dell'aria, con misure che interessano tutti i settori responsabili dell'immissione in aria di sostanze inquinanti nei loro territori, non solo dal settore dei trasporti; basta immaginare la Pianura padana. Con questa norma il Governo ha introdotto l'obbligo per le suddette Regioni di riesaminare i contenuti degli strumenti di pianificazione adottati e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di quantificare l'effettivo contributo alla riduzione delle emissioni di PM10 e ossidi di azoto delle diverse misure ad oggi poste in essere, ivi comprese quelle attuative del predetto accordo e del PNNR. Nelle more degli esiti di tali valutazioni, la norma consente ragionevolmente alle Regioni interessate di disporre la limitazione della circolazione stradale per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. In base alla disposizione, inoltre, la limitazione viene consentita solamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, come è anche previsto dall'accordo di programma del 2017, sopra richiamato. È necessario evidenziare come tali scadenze consentano di tenere in considerazione anche le criticità legate all'indisponibilità dei materiali necessari alla produzione di batterie di veicoli elettrici, per consentire ovviamente la sostituzione dei veicoli euro 5, senza però impattare sulle tempistiche necessarie al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del pacchetto UE «Pronti per il 55 per cento» di riduzione dell'uso di combustibili fossili nei trasporti, che - si ricorda - richiedono inoltre la realizzazione di adeguate infrastrutture per la ricarica o il rifornimento dei veicoli elettrici o alimentati con combustibili alternativi. L'intervento del Governo quindi rappresenta un supporto alle Regioni nel raggiungimento di tali obiettivi, evitando di creare un danno economico e sociale enorme, che il blocco avrebbe causato non solo per i territori coinvolti, ma per l'Italia intera. Con questa norma il Governo intende valorizzare altresì gli effetti delle tante misure messe in campo in questi anni grazie agli investimenti nazionali e alle misure del PNRR, in particolare quelle di efficientamento energetico, considerato che l'inquinamento in Pianura padana non è generato unicamente dal traffico veicolare. È quindi necessario che il Governo continui a portare avanti in modo serio, pragmatico e non ideologico - così come sta facendo - misure efficaci e realistiche per tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute delle persone, evitando ricadute sociali pesanti a carico di migliaia di lavoratori e famiglie. Specificatamente per il settore dei trasporti il Governo e questa maggioranza intendono portare avanti misure ragionevoli per il miglioramento della qualità dell'aria. Ricordiamo in particolare il sostegno nell'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale e il sostegno alle imprese per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. il provvedimento oggi in discussione riguarda la qualità dell'aria e prevede, in primo luogo, che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, ad avviare i piani di qualità dell'aria. A tale riguardo le suddette Regioni possono modificare, se necessario, i provvedimenti attuativi. Questo alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli euro 5 previsto in questo provvedimento. Comprendiamo bene che il Governo aveva premura di intervenire sulla questione. Tuttavia ciò non legittima, né giustifica il solito ricorso dell'Esecutivo a tempi oltremodo stringenti. Per dirla con una metafora calcistica, il Governo si muove ancora una volta in zona Cesarini, il che non consente un'analisi ragionata del decreto-legge in conversione e svilisce, ancora una volta, il ruolo, il lavoro e la dignità parlamentare. Lo abbiamo visto in questo anno di legislatura, lo abbiamo visto la scorsa settimana, riferito alla NADEF, e lo leggiamo dai giornali, già riferito alla prossima manovra di bilancio, dove ci viene spiegato che il Parlamento verrà totalmente messo fuori dalla discussione parlamentare ed emendativa, come la Costituzione vorrebbe. Il Parlamento non può essere organo di ratifica delle decisioni del Governo, spesso avulse da una visione d'insieme e, come in questo caso, viziate da pesanti ritardi dell'Esecutivo, tra l'altro su un tema di primaria importanza, che riguarda la sostenibilità e la transizione *green*, così come la salute degli italiani e l'economia in generale. Nello specifico, la corsa del Governo all'ultimo minuto è dettata dal fatto che nei confronti dell'Italia pendono tre gravi procedure di infrazione. La Commissione europea ha ritenuto di avviarle per cattiva applicazione da parte dell'Italia della direttiva dell'Unione sulla qualità dell'aria. quella relativa al superamento sistematico e continuo dei valori limite di micro particelle PM10 in zone e agglomerati italiani, determinanti da parte dell'Italia, ha dato luogo ad una sentenza della Corte di giustizia europea, che ha accertato la violazione della direttiva, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Di conseguenza, la prospettiva all'orizzonte è, in caso di protratta inerzia, il pagamento di elevate sanzioni da parte dell'Italia. Ancora un'altra procedura di infrazione ha prodotto una specifica sentenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per la violazione della medesima direttiva, rilevando un analogo superamento del valore limite del biossido di azoto. Ancora, il 30 ottobre del 2020 la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione, invitando l'Italia a conformarsi a conformarsi alle prescrizioni della direttiva europea sulla qualità dell'aria. Il richiamo, in questo caso, riguarda il particolato, ossia il cosiddetto PM2,5. Secondo la Commissione, i dati disponibili per l'Italia dimostrano che il valore per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città italiane, soprattutto della valle del Po. ci saremmo aspettati che in questo provvedimento vi fosse un ulteriore incremento delle risorse disponibili, in un'ottica di maggiore e più convinta conformità dell'Italia agli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti previsti a livello sovranazionale e internazionale. La maggioranza potrebbe obiettare che le risorse sono già sufficienti, dati gli incrementi finora avvenuti. Sarebbe, però, una scusa vana. Questa era, infatti, l'occasione per dimostrare una visione matura sui grandi temi dell'ambiente e della sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Purtroppo, invece, il Governo ha utilizzato questa occasione soltanto per allentare l'attenzione e l'attuazione, da parte della Commissione europea, e per evitare sanzioni onerose alla luce delle ricordate sentenze della Corte di giustizia. Del resto, non è una novità che questo Governo voglia mantenersi disallineato rispetto a molti impegni vincolanti nella sede europea. Specie in ordine alla sostenibilità ambientale, il Governo mantiene e continua una intolleranza plateale, che non di rado assume le forme di populismo compiaciuto perpetrato da esponenti della propria maggioranza. *(Applausi)*. Ancora, al comma 2 dell'articolo 1 di questo decreto, dispone che, nelle more dell'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria previsto dal comma precedente, le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale per le autovetture e per i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, alimentate con il *diesel* di categoria euro 5, esclusivamente a partire dal 1° ottobre 2024. In termini più chiari, in questo provvedimento il Governo non è andato non è andato incontro alle aziende, non ha provato ad aiutarle rinunciando totalmente a perseguire politiche di sostenibilità ambientale, che sono strettamente correlate alla sostenibilità economica e sociale. Il Governo, infatti, si limita a misure puramente temporali. Tuttavia, l'Esecutivo non spinge e non aiuta le imprese a cambiare, per esempio, le flotte dei mezzi di trasporto preposti alla logistica; non le aiuta, cioè, a passare ai veicoli elettrici, che ancora oggi hanno uno svantaggio oggettivamente innegabile, rappresentato soprattutto dagli elevati costi di acquisto. Nell'ottica di sostenere le imprese, anche nella competitività e nella creazione di valore dentro il modello di *business* votato alla sostenibilità, il Governo poteva introdurre importanti misure proprio in questo provvedimento. Poteva, cioè, sforzarsi di incentivare le imprese a sostituire le loro flotte con veicoli elettrici. Purtroppo, dobbiamo prendere atto che questo è un Governo sospettoso sulla transizione verde in atto. Sarebbe troppo, per questo Governo ragionare, in prospettiva di *green logistic*. Voglio appena ricordare che il traffico generato dal trasporto merci rappresenta tra il 20 e il 30 per cento dei chilometri percorsi dai veicoli nelle aree urbane e fra il 16 e il 50 per cento dell'inquinamento atmosferico derivante da tutti i tipi di trasporto. ancora una volta il Governo conferma un approccio superficiale, ambiguo e perfino ostile rispetto alla transizione *green* e, più in generale, alle dimensioni della sostenibilità, che invece sono i pilastri su cui dobbiamo costruire e su cui va costruito, all'interno dell'Europa, un futuro migliore per le nuove generazioni. E dico al Governo di opportunità, di equità, di diritti certi, di stabilità ambientale, economica e sociale. Tutto questo, in questo decreto non c'è. Anche questa volta, avete perso un'occasione.

il provvedimento in esame fa riferimento all'attuazione di due sentenze della Corte di giustizia europea, una del 2020 e una del 2022, in materia di inquinamento ambientale, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento da particolato (il PM10) e il biossido di azoto.

insieme hanno consentito di migliorare il testo e di ragionare fino in fondo in Commissione sui contenuti di questo decreto. prevede, per le Regioni interessate in particolar modo dalla sentenza citata (quindi Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) l'obbligo di definire gli strumenti di pianificazione adottati e i relativi provvedimenti attuativi.

senatori dell'opposizione, questo termine è un atto di buon senso perché è finalizzato alla possibilità di mettere in campo strumenti utili a far coesistere la limitazione stessa con le esigenze dei cittadini - anche queste molto importanti - di esercitare un preminente diritto sociale e civile, quindi di rango costituzionale, che è quello alla mobilità è un presupposto, quello di potersi muovere, per poter lavorare, per poter accompagnare un figlio a scuola oppure per un ragazzo andare a scuola o all'università. È in definitiva un principio di libertà. Alla stessa logica risponde l'aver posto un termine iniziale all'l ottobre 2025 per inserire questi provvedimenti in un quadro complessivo di pianificazione. Infatti non si può limitare la circolazione, seppure per meritevoli ragioni - che noi condividiamo e che la Corte europea ha sancito - di tutela della salute, senza garantire ad esempio che per i mezzi elettrici siano disposte ed organizzate le colonnine di ricarica, che sia organizzato anche un sistema di calmierazione del mercato dell'elettrico, che oggi è oggettivamente inaccessibile alla maggior parte del popolo italiano da un punto di vista banalmente reddituale. È necessario mettere in campo questi strumenti e questi interventi ed il termine che viene messo in campo ha questa finalità. È importante in questo senso anche il fatto che la norma abbia fatto riferimento alla necessità di accompagnare questi provvedimenti con la verifica dell'esistenza di un adeguato livello di trasporto pubblico locale. Questo principio per noi di Fratelli Italia è talmente importante ed è a noi così tanto caro che abbiamo presentato proprio qui in Senato un disegno di legge a prima firma della collega Mennuni che lo pone come principio essenziale della pianificazione degli interventi sul territorio, compresi ovviamente quelli di limitazione del trasporto privato, anche da parte degli enti locali. Una proposta che è nata empiricamente dalla situazione della capitale, nella quale l'amministrazione PD - lo dico anche ai colleghi del Partito Democratico - ha pensato ad un sistema di limitazione, che tra l'altro ha determinato proteste a tutti i livelli nel territorio della capitale, che non tiene minimamente conto della drammatica situazione del trasporto pubblico della capitale stessa, certamente non degno della capitale d'Italia. Di recente abbiamo stanziato, come Governo, risorse per il trasporto pubblico della Capitale, per Roma Metropolitane, quindi consigliamo magari al sindaco Gualtieri di utilizzare le risorse che il Governo Meloni mette a disposizione o a blocchi della circolazione per i veicoli privati che metterebbero semplicemente in ginocchio la gente per bene, la gente che la mattina si alza per andare a lavorare. Tornando al decreto-legge in esame, questo principio, volto ad una coesistenza tra diritto alla salute e quello alla mobilità, viene affermato anche attraverso interventi proattivi, come l'emendamento del Governo che stanzia fondi per il turismo ecosostenibile. Tanti altri buoni e buoni e sani comportamenti, compreso l'utilizzo delle tecnologie, si possono mettere in campo; pensiamo alla captazione del PM10, anche nel settore edilizio, e a quanto si può realizzare da questo punto di vista Più in generale, si tratta di mettere da parte, con buona pace di chi le continua a portare avanti astrattamente, visioni integraliste che creano fratture sociali e guerre tra poveri, affermando il principio della necessaria coesistenza tra sostenibilità ambientale,

che è affermato anche in un emendamento di Fratelli d'Italia approvato in Commissione. Tale misura, rispetto a questi provvedimenti di limitazione, fa salvi anche i mezzi che utilizzino dei biocarburanti.

da utilizzare, lavorando ad una transizione ecologica che sia davvero tale e che non azzeri il nostro sistema industriale, ma lo accompagni semmai ad una ridefinizione in chiave sostenibile.

noi preferiamo affidarci all'eresia, che oggi sembra diventata tale, del buon senso e del pragmatismo *(Applausi)*, abbinando la difesa dell'ambiente a quella dei nostri interessi nazionali. Nella vostra visione le due cose sono in contrasto; sono abbinate e questo provvedimento rappresenta esattamente questa sintesi e questa idea.